Grazie

sia in Paesi dello scacchiere mediorientale hanno evidenziato l'innalzamento della minaccia terroristica di matrice jihadista che, presentandosi in forme spesso nuove e di inusitata violenza, costituisce una gravissima insidia per la sicurezza interna ed è fattore di instabilità per Stati - penso a quelli del Nord Africa o anche del vicino Oriente - che versano in complesse e talvolta drammatiche situazioni politiche e sociali. La lotta al terrorismo richiede una strategia complessiva per dare una risposta efficace a una minaccia seria e di notevole entità. Sono ovvie, dunque, la necessità e l'urgenza di predisporre un insieme di norme che, a vari livelli, si preoccupi di rispondere alle esigenze di sicurezza della collettività, a fronte di fenomeni terroristici che, facendoci d'improvviso precipitare nella barbarie, sono drammaticamente assurti agli onori delle cronache. In tale contesto diventa indifferibile rafforzare il quadro normativo vigente, introducendo misure capaci di prevenire il radicamento di tali organizzazioni e di attuare più stringenti controlli sui mezzi e sui materiali che potrebbero essere impiegati per il compimento degli attentati. I fatti di Bari e di Milano, dove due persone sono state fermate con l'accusa di far parte di una cellula terroristica legata allo Stato islamico e ad Al Qaeda e che - secondo gli investigatori - erano pronti a fare attentati in centri commerciali, porti e aeroporti, mostrano un'evidenza che da mesi cerchiamo di porre all'ordine del giorno di una politica italiana che si è emozionata dopo gli atroci attentati di Parigi e Bruxelles, ma poi ha come rimosso il rischio terrorismo. L'Occidente in generale sta sottovalutando la sfida. Cos'altro serve dopo le due torri, dopo Londra, dopo Madrid, dopo Copenaghen, dopo «Charlie Hebdo», dopo il museo Bardo, dopo l'aereo in Egitto, dopo Parigi nel novembre scorso, dopo Bruxelles, per per comprendere che,da ormai quasi quindici anni, il mostro del terrorismo islamista ha scelto la carta degli attacchi indiscriminati su vittime civili? È inutile farsi illusioni. L'Italia è purtroppo un possibile bersaglio, come la propaganda dell'ISIS ripete a chiare lettere. Non possiamo più attendere. Occorre, in particolare, un rafforzamento della missione militare internazionale anti-ISIS per non lasciare Stati falliti e spazi vuoti, dalla Siria alla Libia, dove l'ISIS possa muoversi, prosperare e pianificare. Nel nostro Paese, poi, dobbiamo chiudere immediatamente le moschee irregolari e ogni luogo di culto irregolare e senza controlli, permettendo l'apertura solo di moschee e luoghi di culto autorizzati e controllati. Serve un sistematico controllo del territorio rispetto al fenomeno dei centri di aggregazione clandestini. Nel resto d'Europa bisogna convincere le autorità nazionali ed europee a riguadagnare alla legalità le aree di territorio lasciate, in nome di un multiculturalismo fallimentare e già

Semmai il dato negativo, il punto dolente è che ci sono voluti anni perché il Governo di centrosinistra attualmente in carica - o prevalentemente di sinistra, più correttamente - portasse in Aula la ratifica di questi provvedimenti. Sono passati sei anni e solo oggi si avverte la necessità di provvedere alla ratifica. Ma quel che è peggio è che, mentre ratifichiamo ciò che l'Europa e gli altri Stati europei hanno concordato, rimane assolutamente latitante il Governo italiano per tutto ciò che avviene in Italia. Noi consideriamo la difesa del cittadino sotto l'aspetto della sicurezza interna e internazionale contro il terrorismo, ma anche contro la malavita, una priorità. Consideriamo, anzi, che la sicurezza sia una precondizione di libertà. Senza una volontà politica di contrasto al terrorismo, di contrasto alla criminalità, non vi può essere il libero esercizio di tutte le libertà garantite dalla Costituzione. Non vi può essere la serenità nei trasporti, nei trasferimenti. Non vi può essere la serenità dei genitori nei confronti del figlio che prende la metropolitana per andare a scuola. Non vi può essere la serenità di chi svolge un'attività lavorativa che potrebbe essere minata dal terrorismo e da varie forme di criminalità. In sostanza, non è un'invenzione nostra il termine «sicurezza» interna o internazionale, non è un fatto propagandistico. Qualche volta ho sentito dire: «C'è chi soffia nel fuoco». Ci sembra che ci sia, invece, chi il fuoco fa finta di non vedere a costo di bruciare la libertà dei cittadini. È per questo che votiamo a favore delle ratifiche in esame, mantenendo tutta la nostra critica nei confronti dell'inadeguatezza del Governo a dare risposte su questo terreno.

il pericolo rappresentato dal terrorismo è diventato ancora più insidioso: non solo non è venuto meno, ma ha dato la dimostrazione di poter essere particolarmente insidioso.

pericolose. La Lega Nord non potrà esimersi dal votare a favore delle ratifiche in esame, anche se non possiamo che sottolineare che, probabilmente, si poteva approfittare della circostanza per irrigidire ulteriormente le nostre norme interne

di controllo del territorio. Nonostante queste considerazioni, noi ribadiamo il voto favorevole di tutto il Gruppo della Lega Nord

giunge in Senato, nel Parlamento italiano, con un notevolissimo ritardo. Vi è una evidente contraddizione tra convenzioni e trattati che intervengono

di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; *c*) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo

si è giunti a ratificare trattati e convenzioni. È sorto qualche problema - come abbiamo rilevato nelle sedute precedenti - relativamente a qualche emendamento. Mi riferisco

che si andava a tipizzare il concorso esterno in associazione terroristica e si lasciava quel vuoto del concorso esterno in associazione mafiosa, con ciò determinando, in qualche modo, qualche perplessità su quelle sentenze di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, che vengono sorrette, fondate e motivate sulla base di una derivazione giurisprudenziale. L'argomento non è interessante, per la verità, e - a mio avviso - non è neanche fondato, in considerazione del fatto che, se vi è una norma tipizzata di concorso esterno in associazione terroristica, ben può, in altri casi,

Grazie

dell'armoniosità del sistema penale sotto il profilo sanzionatorio del nostro codice. Come opportunamente sosteneva il senatore Giovanardi quando abbiamo discusso quell'emendamento, non è allora immaginabile condannare una persona che detiene ordigni

Ora vorrei fare soltanto una precisazione sul punto finale: poiché la stampa si è lasciata andare alle considerazioni più svariate, parlando addirittura di pizzini, vorrei chiarire una volta e per sempre in quest'Aula che

Noi non offriamo i numeri. L'ho già detto in altra occasione: noi offriamo contributi di modesta intelligenza e preparazione, ma semplicemente contributi. E li chiamo modesti soltanto perché io sono un uomo modesto, presidente Calderoli, ma tanto modesti, per la verità, non sono. Noi offriamo Noi offriamo questo alla maggioranza. Non siamo nelle condizioni di poter offrire altro, perché in quest'Aula ragioniamo innanzitutto sotto il profilo tecnico e quell'emendamento

un parere favorevole a quell'emendamento. E mi stupisce anche che, sotto il profilo squisitamente politico dell'andamento dei lavori dell'Aula, non si siano resi conto che quell'emendamento sarebbe stato Per quanto riguarda l'intervento del presidente Zanda e il suo riferimento alla Commissione giustizia, noi in quella sede lavoriamo e ci confrontiamo e questo tema era stato trattato e discusso. Ma quando il Governo si impunta su determinate posizioni, non consentendo il confronto all'interno della Commissione, questi poi sono i risultati. La colpa non può essere attribuita né alla Commissione giustizia che lavora e lavora bene,

di dover votare qualcosa che non condividono. La colpa credo sia da attribuire all'atteggiamento arrogante, ottuso in alcuni momenti, del Governo, un Governo che noi continuiamo

in particolar modo quelle di natura squisitamente tecnica. Ciò detto, concludo dicendo che così come sistemato, con l'approvazione degli emendamenti Caliendo 4.10 e 4.12, il provvedimento è da noi

pericoloso, o quanto meno ci ha dato una sensazione di pericolosità anche nel compiere atti normali come prendere una metropolitana o stare in luoghi pieni di gente. Era quello che i terroristi speravano di ottenere. Probabilmente speravano di ottenere anche una risposta securitaria, una risposta a muso duro da parte delle società occidentali che attaccavano, per poter poi impiegare tale risposta quale ulteriore motivazione per combattere contro di noi, contro quelli che loro chiamano i nuovi crociati.

Riteniamo però che questo tipo di risposta, tutta affidata a norme penali o a riduzioni della libertà dei cittadini non sia giusta perché

piena di esplosivo e di farsi - attenzione «farsi» - esplodere in mezzo alla folla, l'inasprimento delle pene

morendo, di finire in paradiso e di essere premiato moltissime volte, sicuramente insieme alla sua famiglia. Quello a cui tutta la società occidentale dovrebbe accedere come tentativo di soluzione e come cura del problema è il prosciugamento delle coltivazioni di odio che nei Paesi del Medio Oriente sono state, negli ultimi decenni, fortemente abbeverate, fortemente concimate da interventi inopportuni, ingiusti e ingiustificabili da parte dell'Occidente. Penso a quello che è successo in Iraq; penso al modo in cui la comunità internazionale sta aiutando i siriani: bombardandoli; penso al modo in cui il sistema occidentale sta respingendo uomini, donne e bambini che tentano di sfuggire alla guerra e alla miseria: appaltando ad altri, per scaricarsi inefficacemente la coscienza, la funzione di gendarmi e di carcerieri (ad esempio, con l'accordo con la Turchia). Certo, però, dobbiamo provare a mettere in piedi una legislazione che renda difficile ai terroristi attaccare le nostre città e la nostra gente. Tuttavia, per farlo dobbiamo fare attenzione ad evitare, in questo impeto difensivo, difensivo, di rendere possibili altre ingiustizie per riduzione della libertà dei nostri cittadini.

il tipo di reato, il modo in cui questo comportamento possa essere definito reato, per evitare di far male volendo far bene. Per questi motivi, per il fatto che non ci dobbiamo e non ci possiamo nascondere dietro norme repressive

Il punto è che la lotta al terrorismo, quella vera, noi la potremmo fare laddove riuscissimo, ad esempio, a fare una seria legislazione e un serio controllo sul traffico d'armi. d'armi. Ho visto molte vignette che sono estremamente esplicative da questo punto di vista: noi esportiamo armi e, assieme al petrolio, importiamo terroristi. Se l'Occidente capirà questo tipo di meccanismo, allora il terrorismo verrà disseccato lì dove nasce. In chiusura di questo intervento, voglio dare atto al relatore, senatore Lo Giudice, di aver operato in modo diverso rispetto alla norma e di avere specificamente motivato i propri pareri sugli emendamenti. È un segno di

Signor Presidente, ci apprestiamo a votare il disegno di legge in esame che dovrà disporre la ratifica e l'attuazione di cinque trattati e convenzioni internazionali in materia di terrorismo, di contrasto

fare delle considerazioni *a latere.* Infatti, pur non essendo direttamente ed espressamente attinente al contenuto dei trattati e delle disposizioni normative penali che andiamo a introdurre, non possiamo non richiamare anche in questa sede una riflessione più generale sul fatto che il fenomeno terroristico, soprattutto quello di natura mediorientale, nasce e cresce in virtù della situazione geopolitica internazionale e delle politiche politiche che la comunità internazionale (soprattutto da parte di quegli organismi di cui facciamo parte) ha contribuito a creare come situazione generale. Riteniamo quindi che il ruolo dell'Italia per contrastare il terrorismo potrebbe politici concreti, come ad esempio l'attuazione di una immediata moratoria della vendita d'armi a Paesi come, ad esempio, l'Arabia Saudita, che sappiamo utilizza armamenti anche di origine italiana per azioni militari contro le popolazioni civili dello Yemen. L'Italia potrebbe rinegoziare il proprio ruolo nell'ambito della NATO, che ormai, da alleanza difensiva, è diventata un'alleanza troppo spesso di guerra; dovrebbe rivedere l'impianto sanzionatorio contro la Russia, recentemente confermato e prorogato per ulteriori sei mesi. Tutto ciò nell'ambito dell'inquadramento della situazione politica situazione politica italiana negli organismi internazionali. Ciò detto e richiamando la necessità di questo tipo di azione politica nel merito del disegno di legge, tanto più dopo la modifica intervenuta la settimana scorsa con l'approvazione di un emendamento che - come sappiamo - ha aumentato la pena base per un reato molto grave relativo al terrorismo cosiddetto nucleare, il nostro voto sarà favorevole perché, oltre alla necessaria ratifica dei trattati e delle convenzioni, ricordiamo che con il presente disegno di legge si introducono nuovi reati. Con questa modifica del codice penale è previsto il nuovo reato di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, il reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro. Le disposizioni in esame introducono misure di carattere penale volte a contrastare anche le forme di finanziamento alle attività terroristiche basate sull'utilizzo di fondi provenienti da attività lecite, ovvero quelle attività che, pur non avendo un disvalore intrinseco e non essendo quindi - a legislazione vigente - giuridicamente vietate, vietate, per le loro caratteristiche possono però essere utilizzate in modo strumentale dalle organizzazioni terroristiche. Positivo è il nostro giudizio anche sulla norma che prevede, in caso di condanna o anche di patteggiamento per questi reati, sia disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato; tale confisca è prevista anche per equivalente. Altrettanto da salutare positivamente sono le nuove disposizioni normative che puniscono gli atti del cosiddetto terrorismo nucleare.

Forse, in tutto il dispositivo normativo introdotto, quello che ha destato particolarmente il nostro interesse è quanto previsto e disposto dall'articolo 5 del disegno di legge, che stabilisce che il personale dei Servizi d'informazione e sicurezza interna e esterna (quindi l'AISI, l'AISE analogamente alla polizia giudiziaria, è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione a una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei confronti degli agenti dei

previste dalla legge come reato legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso

qualora fossero volte contro l'amministrazione della giustizia, come, ad esempio, in ipotesi di depistaggio. Con tutti questi limiti, ancora una volta, sperimentiamo che nel nostro ordinamento esiste già la figura dell'agente provocatore. Ricordo, ancora una volta, che tale figura è da distinguere dall'agente sotto copertura nei termini tecnici o paratecnici in cui spesso ci riferiamo a queste figure. L'agente sotto copertura è colui che non pone in essere condotte volte alla commissione di reati, ma che si infiltra nelle organizzazioni.

che tale figura non è compatibile, che occorre tempo. Il Governo ha approvato un ordine del giorno in materia di reati contro la pubblica amministrazione con riferimento all'agente sotto copertura, ma «scopriamo» che da quasi un decennio è vigente nel nostro ordinamento, seppur con i limiti di cui ho parlato, una figura ben più forte: quella dell'agente provocatore. Nel votare a favore di questo disegno di legge, che nel campo specifico estende la non punibilità degli agenti provocatori dei servizi anche ai nuovi reati che stiamo introducendo, allora richiamare questo principio affinché valga nella prossima occasione in cui si parlerà di contrasto alla corruzione, e sentiremo delle giustificazioni apparentemente ragionevoli che contrastano con la possibilità di poter introdurre in astratto una figura dell'agente provocatore scriminato nel nostro ordinamento. Questa figura c'è già e ogni giustificazione giuridica o paragiuridica in tal senso sarà sconfessata dalla realtà normativa oggi in vigore.

siamo d'accordo per la ratifica della Convenzione e saremmo stati d'accordo anche su tutte le norme che riguardavano la prevenzione. Avevamo presentato degli emendamenti solo di natura tecnica. Di questi emendamenti, come sapete, due sono stati accolti, ma noi dobbiamo astenerci dal votare questo provvedimento perché

Quando emerge nel dibattito, in Commissione o in Assemblea, la possibilità di una diversa interpretazione di una diversa applicazione, è compito del legislatore trovare delle soluzioni che evitino quell'applicazione distorta o dubbia da parte dei giudici.

il nostro emendamento aveva sollevato e illustrato il collega senatore Palma, poneva un problema in relazione al primo articolo, in particolare per quanto concerne l'applicazione del concorso esterno.

Tutti i giuristi scrivono che se la norma non è chiara, non c'è possibilità di avere certezza dell'interpretazione. Badate che tra le cause della criminalità la non certezza del diritto, che è fondata anche sulla prevedibilità delle decisioni dei giudici. Ciascun cittadino dovrebbe avere la possibilità di prevedere come il giudice applicherà la norma. Solo così i principi fondamentali in materia di obbligatorietà e di uguaglianza dei cittadini potranno avere una concreta attuazione. Queste sono le ragioni che ci portano ad astenerci in questa votazione, pur condividendo le ragioni dell'approvazione della ratifica e delle norme ad essa sottese. colleghi, nel nostro Paese c'è piena consapevolezza che la lotta al terrorismo è una sfida drammatica.

Abbiamo compreso che con il terrorismo non si scherza, che sottovalutare il fenomeno è un errore grave. Abbiamo anche capito che è necessario unire il Paese e dotare il nostro sistema di strumenti adeguati a colpire l'organizzazione terroristica. al complesso culturale e sociale della partecipazione e della capacità di intervenire, sia sul piano preventivo che repressivo, abbiamo vinto e abbiamo superato una stagione difficilissima, segnata da omicidi, da barbari assassini, ma anche dalla capacità di reazione democratica, corale, forte e qualificata della nostra democrazia. Adesso, colleghi, ci troviamo di fronte ad una nuova fase della lotta al terrorismo; un terrorismo globale che è in grado di intervenire sui nostri territori, ma al contempo anche in teatri diversi, lontano da noi. È il terrorismo religioso, quello guidato dall'ISIS, quel terrorismo radicale, che ha costruito una fitta rete di relazioni, in grado di utilizzare le moderne tecnologie, capace di intervenire nel disagio sociale e, in modo perverso, raccogliere consenso e motivare all'azione; in grado di strutturarsi non solo a livello organizzativo, diremmo, sul piano penale, associativo, ma anche attivando singole persone, singoli terroristi all'azione anche terrificante, come abbiamo potuto constatare sia a Parigi, che a Bruxelles, che a Tunisi e nelle diverse azioni che hanno condotto in quella sorta di *via crucis* che tutti abbiamo imparato, ahimè, drammaticamente, a conoscere. Cari colleghi, abbiamo anche capito che di fronte a questo terrorismo, territoriale e globale allo stesso tempo, capace di agire sulle moderne tecnologie e capace di affondare il colpo in modo devastante in grado di frequentare i salotti dell'alta finanza e, contemporaneamente, di inserirsi all'interno del disagio sociale più peculiare nei nostri quartieri, nei quartieri delle città d'Europa,

quella repressiva, che trattiamo oggi, ma anche quella culturale, che non vorrei fosse mai trascurata, sul piano territoriale e globale, con un coordinamento che ha fatto dei passi avanti, che sono però ancora del tutto insufficienti. Ecco perché il nostro Governo sul piano europeo ha chiesto che sul versante dello spazio comune antiterrorismo, così come su quello antimafia, si debba avere più coraggio, più velocità, più comprensione, più integrazione. Cari colleghi, con questo provvedimento immettiamo un altro tassello normativo nel complesso e variegato sistema penale di lotta al terrorismo. Molte nome previste dalle convenzioni internazionali in esame, che ricordo sono ben cinque, sono già presenti nel nostro codice. Alcune sono figlie, come ricordavo prima, della nostra tragica e vincente lotta al terrorismo interno; altre le abbiamo inserite man mano che si agiva contro il nuovo terrorismo. In questo disegno di legge si colpiscono due nuove e importanti fattispecie; si interviene nel delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, al di là che si sia interni all'associazione o si sia partecipi anche attraverso l'istituto giurisprudenziale del concorso esterno.

abbiamo dato anche una nuova risposta e così siamo intervenuti quando si sottraggono beni o denari sottoposti a sequestro. Un altro "buco" che viene finalmente riempito. Si interviene anche quando si è disposta la confisca di cose che servirono o furono destinate a commettere reato e magari, poi, alla fine, non hanno raggiunto questa finalità. Quei beni vengono però sottratti; quei beni sono tolti al terrorismo e recuperati all'azione dello Stato. Cari colleghi,

ed il Governo degli Stati uniti messicani, con allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011. L'Accordo, che si compone di 23 articoli, un preambolo e un allegato, favorisce la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in materia doganale stabilisce l'impegno delle parti a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione per assicurare la corretta applicazione delle rispettive legislazioni e migliorare le azioni di accertamento e repressione delle violazioni. L'Accordo regolamenta le modalità per la comunicazione e lo scambio delle informazioni e descrive la tipologia di informazioni interessate. tra le due autorità doganali, con particolare riferimento alla trasmissione di documenti, con un impegno di speciale sorveglianza su persone e merci che si presume coinvolti in violazioni delle normative doganali. L'Accordo disciplina, inoltre, i casi in cui l'assistenza possa essere rifiutata; fissa i criteri di ripartizione delle spese fra le parti e definisce l'ambito territoriale di applicazione e le ipotesi di risoluzione delle controversie. La stipula dell'Accordo si è resa necessaria per disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali, nel quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le rispettive amministrazioni. L'Accordo potrà consentire di di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali; rafforzare i mezzi di lotta contro la frode; contrastare il traffico illecito degli stupefacenti; agevolare e semplificare le procedure doganali connesse a ogni legittima transazione, rendendo più trasparente l'interscambio commerciale e meno oneroso il compito degli operatori. Il provvedimento regolamenta lo sviluppo dei rapporti diretti ed immediati tra l'Agenzia italiana e l'amministrazione doganale messicana in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'intervento presenta numerosi vantaggi, come quello di regolare in maniera schematica e certa gli interscambi tra i due Paesi, attualmente non disciplinati. I destinatari diretti, cioè le amministrazioni doganali, potranno infatti beneficiare di maggiore cooperazione bilaterale, con i conseguenti effetti positivi sulle attività di prevenzione. Allo stesso modo, i destinatari indiretti, cioè gli operatori economici, beneficeranno di agevolazioni e semplificazioni connesse alle procedure doganali per ogni legittima transazione e di una maggiore trasparenza nelle attività di interscambio commerciale tra i due Paesi. Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli. All'onere economico derivante dal presente Accordo (articolo 3), valutato in 17.800 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, L'Accordo non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

senatore Sangalli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

L'Accordo in discussione regolamenta la cooperazione tecnica e la reciproca assistenza nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico; coinvolge le forze di polizia per la lotta alla criminalità transnazionale ed al terrorismo. La definizione dell'Intesa si è resa necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale in materia di sicurezza ben strutturata e maggiormente corrispondente alle attuali esigenze dei due Paesi, rafforzando le relazioni bilaterali tra l'Italia e l'Angola per lo sviluppo e la tutela di interessi strategici. Nell'Accordo è previsto un riferimento alla cooperazione per l'identificazione e la riammissione di cittadini in posizione irregolare, velocizzando e facilitando l'espulsione dal Paese in cui sosta illegalmente, che ovviamente va nella direzione delle proposte fatte dal Movimento 5 Stelle in tema di flussi migratori. L'Angola, dalla fine della guerra civile nel 2002, grazie ad ambiziosi programmi implementati con l'ausilio di *partner* internazionali, ha saputo entrare nel novero delle economie più dinamiche a livello africano, facendo registrare tassi di crescita a due cifre nell'ultimo decennio. Metà della ricchezza nazionale proviene dal petrolio e da questo dipendono, per la maggior parte, le aspettative di sviluppo di lungo periodo. La produzione dell'oro nero ha conosciuto un autentico *boom* dall'inizio del nuovo millennio, passando da 800.000 barili al giorno agli attuali 1,8 milioni, Il PIL ha avuto una crescita notevole, passando dal 3,4 per cento nel 2003 L'economia angolana è una delle poche a livello mondiale che ha avuto una tale crescita. Il PIL *pro capite* è passato dai 700 dollari nel 2002 a 5.700 dollari quest'anno. L'inflazione, che nel 2002 (anno della prima firma degli accordi di pace) era del 105 per cento, si è ridotta al 7 per cento, e si spera possa ridursi ancora nell'anno in corso. Nonostante ciò, il Paese presenta ancora troppi punti oscuri nel cammino verso una condizione democratica piena: libertà di stampa e di parola ancora troppo limitate, tensioni mai sopite con i gruppi militari protagonisti della guerra civile, corruzione e nepotismo diffusi. È necessario però dare fiducia a questa nuova realtà e appoggiare gli sforzi per un Paese più sicuro. Riteniamo quindi che le politiche di assistenza reciproche di cooperazione tra le polizie importanti per mantenere la stabilità nel Paese e, inoltre, per velocizzare le pratiche di rimpatrio degli angolani illegalmente residenti in Italia. Dichiaro pertanto il nostro voto favorevole.

e la reciproca assistenza nell'azione di contrasto al crimine organizzato transnazionale ed al terrorismo internazionale. I settori di cooperazione previsti dall'Accordo sono, tra gli altri, il traffico illegale di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti

Signor Presidente, nell'anticipare il voto favorevole a questo provvedimento, ricordo solo che in questo Paese effettivamente esistono alcune problematiche che con questo provvedimento vengono risolte. Si tratta di problematiche che riguardano sia l'uno che l'altro Paese.

importante per i traffici internazionali di droga ed un luogo di interesse per le organizzazioni criminali transnazionali. Da lì partono molti scafisti per il traffico di esseri umani. Per detti

Parlamento si occupi maggiormente di queste tematiche e che, soprattutto, lo facciano anche gli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte. Quindi, dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

Ilrelatore facente funzioni, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

non dimentichiamo che l'Armenia è membro del partenariato euro-atlantico, ovvero di quel *forum* di regolare consultazione, coordinamento e dialogo tra la NATO e i suoi *partner* Grazie, accordo si sviluppi e si disciplini la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la cooperazione in materia di sicurezza, la dice lunga, perché sicuramente, se questo fosse stato fatto cento anni fa, non ci sarebbe stata la tremenda sciagura che ha colpito il popolo armeno. l'Accordo che andiamo a ratificare rientra nella categoria di quei patti bilaterali finalizzati a consolidare e aumentare il più possibile la collaborazione militare tra Stati. In poche battute, continuare ad armare il mondo in modo che i conflitti si risolvano sempre con la stessa metodologia, la guerra, assicurando così ai soliti noti di continuare ad arricchirsi (mi riferisco alle industrie belliche), non rientra assolutamente in quell'operazione che l'Italia dovrebbe

Siamo ben consapevoli che, in molte circostanze, gli accordi militari sono assolutamente indispensabili per poter sviluppare relazioni di natura politica e relazioni internazionali adeguate. In questo caso è un accordo di collaborazione con un Paese amico cui forniamo supporto in un'area particolarmente delicata del mondo.

Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012;

Signor Presidente, prima di consegnare la relazione scritta mi conceda due osservazioni:

lei sa quanto io apprezzi il suo modo di presiedere la nostra Aula. Posso capire la fretta, ma questa fretta la notiamo quasi sempre quando si parla di ratifiche di accordi internazionali

Presidente non si innervosisce, è al resto del suo Gruppo che deve rispondere. ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: Il secondo è un Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica delle Filippine dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. Non leggerò tutta la relazione, ma questi accordi spaziano su moltissimi temi. Addirittura quello con l'Iraq, che ha 124 articoli, va dal dialogo politico, alle relazioni commerciali, agli aiuti allo sviluppo, a una serie di ambiti settoriali, dall'ambiente all'energia, dall'istruzione, alla cultura fino ai diritti umani.

Signor Presidente, ha ragione il collega Micheloni: non è un problema di Assemblee parlamentari ma di maggioranza di Governo, che dal 2011 al 2012 è omogenea, uguale

qualche settimana fa, in occasione della precedente infornata di ratifiche, il senatore D'Alì aveva fatto notare che non è opportuno inserire in un solo provvedimento ratifiche di accordi disomogenei. Che c'entra l'accordo con le Filippine con quello con l'Iraq? Mi sembra che entrambi i Paesi abbiano delle specificità e non c'è ragione di votare insieme Le parole del senatore D'Alì, alle quali si sono associati anche altri colleghi, non sono state ascoltate. Vorrei a questo punto ricordare al Governo che la prossima volta che ci sottoporrà

Malan ha fatto un'osservazione circa l'eterogeneità dei provvedimenti di ratifica nell'ambito dello stesso disegno di legge.

che forse l'Italia e l'Europa si dovrebbero porre. Al di là di questo, si tratta di un accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Repubblica delle Filippine noi riteniamo che quando vi siano accordi di cooperazione non vi può che essere un parere favorevole e quindi una sollecitazione a fare

Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare l'Accordo, già approvato dalla Camera dei deputati, di associazione tra l'Unione europea e i sei Paesi dell'America centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), considerati come un'entità regionale integrata. Si tratta di Paesi che dal dicembre del 2003 hanno sottoscritto un Accordo di dialogo politico e di cooperazione con l'Unione europea e che costituiscono una specifica entità regionale integrata chiamata Mercato comune centroamericano, iniziato sin nel 1960. L'Accordo, già ratificato dai sei Paesi interessati, è in linea con l'obiettivo dell'Unione europea di consolidare l'integrazione regionale in altre aree del mondo. L'Accordo è composto, oltre al preambolo, di 363 articoli, 21 allegati, dichiarazioni e un protocollo relativo alla cooperazione culturale. Si rileva, in particolare, la mole dell'Allegato 1 dedicato ai dazi doganali che, da solo, occupa quasi 1.700 pagine. La prima parte (articoli da 1 a 11), dedicata alle disposizioni generali, definisce il quadro istituzionale per la gestione dell'Accordo, prevedendo (articolo 4) la creazione di un Consiglio di associazione, composto dai rappresentanti ministeriali dei Paesi parte. La parte seconda (articoli da 12 a 23) riguarda i profili del dialogo politico tra l'Unione europea e l'America Centrale, tra cui il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (articoli 14 e 15), il terrorismo (articolo 16) e la cooperazione in materia ambientale e fiscale. La terza parte dell'Accordo (articoli da 24 a 76) riguarda i diversi aspetti della cooperazione nel settore della giustizia, della sicurezza e dello sviluppo sociale. È da segnalare anche l'impegno per la riduzione della povertà dell'esclusione sociale, nonché le iniziative nel campo dell'istruzione, della sanità e della protezione dei popoli indigeni (articolo 45). Relativamente alle migrazioni, l'articolo 49 prevede la cooperazione fra le parti sui diversi profili della materia, a partire dallo *status* dei rifugiati e inclusi quelli criminali come la tratta di esseri umani. La quarta parte dell'Accordo (articoli da 77 a 351) è dedicata alla materia del commercio, prevedendo la creazione di una zona di libero scambio (articolo 77), in conformità con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 78), la riduzione degli ostacoli tariffari e non al commercio. La durata del Accordo è illimitata. Il disegno di legge di ratifica, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, si compone di cinque articoli. Gli oneri economici (articolo 3, comma 1) per l'Italia sono valutati in circa 20.160 euro annui a decorrere dal 2016.

b) *Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra

Il secondo testo è il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, finalizzato a promuovere rapporti di collaborazione bilaterale, al momento non regolati da alcun accordo.

questo è un percorso di avvicinamento all'Unione che passa inevitabilmente per la soluzione della questione relativa al suo *status* internazionale e per il progressivo miglioramento miglioramento dei rapporti con la Serbia. Crediamo pertanto che questa sia un ratifica necessaria se non vogliamo fare di questo Stato un luogo dove ci sia

regna la legge del più forte. La guerra fredda con i Paesi confinanti ha allevato generazioni di combattenti ed è stata terreno fertile per la formazione di organizzazioni combattenti prima e di gruppi criminali poi. Il sentimento nazionalista è molto forte e, di conseguenza, è forte il problema delle minoranze serbe che sono state duramente perseguitate e costrette a lasciare la regione. I traffici illegali di armi, droghe, essere umani e parti di essi sono molto attivi. Per quanto riguarda il trattato in oggetto, ribadisco che il Movimento 5 Stelle ritiene fondamentale promuovere utili forme di collaborazione in materia di assistenza giudiziaria penale. Per questi motivi il mio Gruppo appoggerà questi due accordi internazionali, esprimendo un voto favorevole.

I Paesi dell'Unione europea e i Paesi africani che vengono considerati sono ovviamente dei Paesi differenti. In questo caso non stiamo trattando

Convenzione è stata sottoscritta nel 2015 e costituisce il primo accordo bilaterale sullo scambio di informazioni in materia fiscale sottoscritto dal Vaticano con un altro Paese; quindi è importante. Il testo è in linea con il processo, in atto da diversi anni a livello internazionale, di rafforzamento della trasparenza nelle relazioni finanziarie e segue, come molti altri trattati in materia sottoscritti dal nostro Paese, il modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Lo scambio di informazioni riguarda il periodo di imposta a partire dal 1º gennaio 2009.

Il provvedimento è finalizzato ad aggiornare la precedente intesa istitutiva della Forza militare, armonizzandola alle mutate esigenze operative ed addestrative e ai mutamenti nel frattempo intervenuti a livello internazionale, rafforzando la cooperazione militare dei tre Paesi nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea e alla NATO. Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. Chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto

*(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del Movimento 5 Stelle, soprattutto perché questa è l'ennesima prova che dietro fantomatiche operazioni umanitarie Se andiamo a leggere il *memorandum*, emerge che qui si vuol fare una difesa militare, di armi, di addestramenti e schieramenti a fini dissuasivi, che spesso sono attacchi mascherati. Questo significa guerra e per questo motivo il Movimento 5 Stelle voterà convintamente no.

Grazie,